(Segue la verifica del numero legale). Il Senato è in numero legale.

Voglio ricordare in quest’Aula la prematura scomparsa del senatore Massimo Bonavita. Senatore per tre legislature (dal 1994 al 2006), dapprima per il Gruppo dei Progressisti (dal 1994 al 1996), poi rieletto nelle liste dei Democratici di Sinistra nelle successive due legislature (dal 1996 al 2006).

La sua morte rattrista tutti coloro che lo hanno conosciuto, in particolare a Cesena, dove era stato un protagonista della politica cittadina, fin da giovanissimo impegnato nel Movimento studentesco, poi nel PdUP, di seguito nel Partito Comunista per aderire infine al Partito Democratico di Sinistra del quale fu segretario comunale. Conoscevo bene Massimo Bonavita, e avevo avuto modo di collaborare con lui quando, come giovane assessore del Comune di Cesena, dove lui ricopriva l’incarico di vice segretario generale, ci trovammo a lavorare fianco a fianco. Poi divenne senatore, ed ho un ricordo molto vivo degli incontri nei quali ci parlava del suo lavoro in Senato, dove seguiva in particolare i provvedimenti in tema di bilancio e finanze. Viveva da anni negli Stati Uniti, a Minneapolis dove ha fondato un Centro italiano di cultura con il compito di promuovere la lingua e la cultura italiana. Aveva quindi abbandonato ogni impegno diretto ma continuava, in questo modo, ad interessarsi di politica con la sua consueta passione, contribuendo contribuendo a far conoscere ed apprezzare la cultura italiana nel mondo. Voglio esprimere da questi banchi il mio cordoglio ai familiari. Sapevo della sua malattia ma confidavo che riuscisse a sconfiggerla.

raccontando, in un articolo pubblicato lo scorso dicembre, la scoperta della malattia, gli esami, il rapporto con i medici, l’importanza della speranza. Aveva, insomma, voluto condividere la sua esperienza. Credo Credo lo abbia fatto per aiutare altri nella sua situazione, per dire che non bisogna isolarsi, né chiudersi ma affrontare con forza, con la “giusta reazione”, anche una esperienza così difficile e dolorosa. Un invito alla condivisione e alla speranza che costituisce la cifra più profonda e vera di chi, come lui, ha vissuto la politica come un impegno fondato sui valori e sulla volontà di costruire un mondo migliore, un modo di vivere il presente con lo sguardo proiettato al futuro.

l’ho conosciuto perché sono stata una delle migliori perdenti quando lui era già senatore e fu il primo a congratularsi con me. Io fui una spuria qui in Senato

un uomo che ha servito con passione il Senato e il suo territorio. È per questo che lo vogliamo ricordare. Lo vogliamo anche ricordare, signora Presidente, perché il ricordo di un persona che ha servito con passione le istituzioni, anche se molti di noi non lo hanno conosciuto, è importante per non disperdere questa passione, questo modo di stare mezzo alla gente e con la gente, in maniera precisa e puntuale e al fine di servire le persone. Quindi, lo ricordo con estremo affetto e anche con grande rammarico. Conosco molto bene la famiglia e a loro faccio le mie più sentite condoglianze. Le faccio anche al Partito Democratico, perché è stato un uomo del partito e con il partito.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al rimpianto e al ricordo della figura del senatore Bonavita prematuramente scomparso e si associa anche al cordoglio per la famiglia.

che con i loro interventi di ieri hanno certamente arricchito l’esame di un provvedimento del quale tutti riconoscono l’importanza, anche chi lo ha fatto con accenni critici ma - mi è sembrato di cogliere - mossi da un intento costruttivo. La mia replica sarà breve e toccherà alcuni aspetti di tipo generale; so che il Governo si riserverà poi di entrare più nel dettaglio. Parto da un dato che anch’io avevo segnalato ed è stato ripreso da molti: il provvedimento che è al nostro esame ha un iter lungo alle sue spalle, ma lasciatemi sottolineare che questo non significa che sia stato un trascorrere di tempo inutile. Alcune parti più urgenti del disegno di legge quale era in origine sono già in vigore, da tempo, essendo state oggetto di stralcio ed essendo state inserite in altri veicoli normativi, perché l’urgenza lì spingeva l’azione di Governo. Nel corso del tempo parti nuove si sono aggiunte sia nella prima lettura al Senato che alla Camera dei deputati. In ogni caso credo che tutti possano riconoscere che il disegno di legge conserva oggi una sua vera organicità, in parte con differenti caratterizzazioni, in parte conservando molti aspetti dell’impianto originario. Le novità derivano proprio da un maggior approfondimento e da un adattamento al mutato contesto politico e fattuale generale e settoriale. Non sto qui a ribadire - l’ho già fatto ieri in dettaglio - gli ambiti di intervento più importanti del disegno di legge. Lasciatemi però sottolineare una volta di più che sono ambiti di primario rilievo che hanno trovato appoggio e sostegno da parte del vasto mondo dei diretti interessati. Voglio anche citare - perché ne ho preso nota nel corso del dibattito - le problematiche che sono state sollevate, che afferiscono a materie indubbiamente importanti di cui è stata lamentata la non presenza nel disegno di legge. Ma anche qui l’osservazione che voglio fare è che non si tratta di un provvedimento omnibus. I temi che sono stati ricordati sono importanti: chi ha citato le quote latte, chi la concorrenza delle importazioni di riso dall’estero, chi l’agricoltura montana, chi l’istruzione agraria, chi le emergenze fitosanitarie e la ricerca scientifica, chi la criminalità agroambientale, chi i pesticidi, chi gli squilibri nella filiera agroalimentare, chi la tutela in generale del patrimonio agroalimentare italiano o l’importante tema dell’imprenditoria femminile in

agricoltura - che di alcune di queste tematiche la Commissione agricoltura già si sta occupando da tempo, con solerzia e con diligenza. quindi, in grado di proporre all’Assemblea interventi specifici su questi temi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Altri temi sono all’ordine del giorno o sono nei nostri progetti di intervento. Credo, dunque, che si possa dire che, complessivamente, il Senato, la sua Commissione e il Governo stanno cercando di delineare, nel corso di questa legislatura, un intervento organico sul complesso delle tematiche che riguardano il comparto primario.

Questo provvedimento rappresenta - lo dicevo già ieri - per certi versi un punto di arrivo, per altri un punto di partenza. Consegniamo nelle mani del Governo importanti deleghe e ci auguriamo che ci sia, da parte del Governo, un’azione sollecita affinché queste deleghe, una volta attuate, diano ulteriore certezza normativa al sistema. Peraltro, le disposizioni immediatamente precettive sono, per certi versi, ancora più numerose e importanti delle deleghe e consentiranno con immediatezza semplificazioni normative. Sottolineo questo tema: di semplificazioni il Parlamento e l’opinione pubblica dibattono da troppo da troppo tempo, ma le semplificazioni contenute in questo provvedimento rispondono ad importanti richieste e faciliteranno la vita e il lavoro degli addetti. Ci sono misure di sostegno in settori produttivi, misure di incontro tra domanda e offerta di terreni agricoli; interveniamo sulla funzionalità delle attività agricole mediante i contratti di rete, di rete, il contrasto alle infrazioni in materia di pesca e acquacoltura e al bracconaggio ittico nelle acque interne. Mai come in questa legislatura

oltre importanti profili di competenze in leggi più ampie, primo tra tutti il decreto-legge competitività. Ancora una volta, in questo campo i dati economici ci danno ragione. I dati economici confermano un andamento positivo del comparto agricolo; certo, non esente da criticità, ma il segno complessivo è nettamente positivo. quindi, di una tendenza che deve essere sostenuta e consolidata, perché può rendere ancora più importante l’azione dei nostri concittadini impegnati in questo settore; e questo nonostante non manchino le difficoltà, che provengono da cause naturali (le numerose calamità) o sono di tipo politico (penso all’embargo russo e alla concorrenza sempre sleale che dobbiamo verificare sui mercati esteri). A queste sfide stiamo rispondendo - e vogliamo sempre più rispondere - con la tutela delle eccellenze e delle qualità che rendono i nostri prodotti agroalimentari i più noti nel mondo.

Il disegno di legge che quest’Assemblea si appresta a votare per la seconda volta rappresenta, come è stato ricordato, il frutto di un ampio ed importante lavoro, condiviso dal Governo e dal Parlamento, che è durato oltre due anni: questo è stato il primo motivo di grande critica ed è naturale e per certi versi anche giusto che sia così. Certamente il provvedimento ha avuto un iter troppo ha detto il ministro Martina nei giorni passati, come è stato giustamente ricordato. Vi è, tuttavia, un punto che vorrei sottolineare alla vostra attenzione,

in questo o in altri provvedimenti ed è diventato legge dello Stato, parte integrante della strategia del nostro Esecutivo per il comparto agricolo: questo è un passaggio che considero davvero importante nella relazione fattiva con il Parlamento. Non vi è soltanto la necessità di approvare delle leggi, ma anche quella di affrontare dei temi e di far sì che i cittadini e le nostre imprese abbiano risposte rispetto alle questioni che oggi vengono poste sul tappeto in tale logica che ci siamo mossi in questi due anni. Ha ragione chi ha notato la perdita, per alcuni versi, di un disegno unitario coerente in alcune parti del provvedimento in esame. Chiaramente nel tempo vi sono stati

nei mesi e negli anni passati, ci accorgiamo che quella coerenza che parzialmente nel testo in esame è stata persa, non è stata persa nel disegno complessivo.

Come giustamente è stato rilevato dai colleghi di maggioranza (penso al senatore Ruta), noi abbiamo l’orgoglio di avere portato a casa in questi anni - e non è soltanto un orgoglio di parte - un progetto unitario rispetto alla nostra agricoltura. 6 Luglio 2016 questo Parlamento imprimerà una svolta importante, veramente molto importante, all’intero comparto agricolo, in linea con tutti i provvedimenti già compiuti compiuti e con quelli in itinere nelle Camere, volti a rafforzare un settore che rappresenta un’indiscussa eccellenza per il nostro Paese.

Possiamo tutti quanti (e io peraltro sono tra coloro che lo fanno più spesso) guardare al bicchiere mezzo vuoto, cioè non essere assertori di una visione ottimistica a tutto campo, non dimentichiamoci i dati assoluti,

la crescita dell’occupazione in agricoltura del 2,2 per cento (e continua a farlo, perché è cresciuta anche nei due anni precedenti) ci dicono che non stiamo sbagliando la strada. Potete spronarci finché volete, fate bene ed è giusto che sia così affinché facciamo di più e meglio; su questo siamo d’accordo, ma non stiamo sbagliando la strada: la strada è quella giusta e sta dando i risultati sperati; anzi, oggi alcuni indicatori sono migliori di quanto ci si potesse attendere. Stiamo parlando di valore aggiunto in agricoltura e non soltanto di crescita dell’export agroalimentare, che naturalmente ci inorgoglisce moltissimo e di cui andiamo fieri, ma che può rappresentare una svolta e una crescita più per l’agroindustria che per il comparto primario.

in questo Paese. È un segnale di grande attenzione specifica ai singoli settori, al settore lattiero-caseario e alle varie crisi manifestatesi, rispetto alle quali non stiamo fermi e continueremo a lavorare perché sappiamo essere priorità per il Paese.

Rapidamente mi soffermo su alcune indicazioni di questo provvedimento, ricordando soltanto quelli più qualificanti, a mio parere. Innanzitutto vi è la fondamentale opera di semplificazione sia normativa che burocratica prevista dal disegno di legge,

non passare per una riorganizzazione improntata all’efficientamento dei principali interlocutori degli agricoltori, ovvero i nostri enti, per i quali abbiamo avviato da tempo una drastica opera di ripensamento, che intendiamo continuare al fine di garantire un migliore servizio, con un più razionale impiego delle risorse pubbliche. Vi sono, infine, attesi interventi per alcuni specifici settori, anche a tutela delle realtà più piccole e fragili della nostra agricoltura, ma non per questo meno pregiate per qualità,

del Paese e nel confronto con i parlamentari l’elemento qualificante dell’azione di Governo. condotto da questo Senato per oltre un anno, e dopo un secondo esame portato avanti dalla Camera dei deputati per quasi un ulteriore anno, che certamente hanno contribuito ad arricchire e a migliorare il provvedimento, ritengo che il disegno di legge sia maturo per la definitiva approvazione da parte del Parlamento. Per tale ragione, dico già da ora che il Governo ritiene di dovere esprimere un parere contrario su tutti gli emendamenti, garantendo comunque (ci tengo a sottolinearlo per tutti i colleghi, ma lo dico in particolare a chi aveva chiesto una particolare attenzione rispetto alle questioni sollevate), attraverso una volontà di leale collaborazione con il Parlamento, la massima considerazione delle questioni messe in luce da questa Assemblea, in particolare attraverso gli ordini del giorno, soprattutto riguardo al riordino della disciplina dei consorzi e su altre materie che sappiamo essere alla vostra attenzione. Non possiamo più attendere questa fondamentale opera di rilancio del settore agricolo, e oggi, credo, insieme, colleghi - spero con una convergenza ampia di tutti voi possiamo costruire il futuro di un comparto primario in tutti i sensi per il Paese. Non mancheranno occasioni per confrontarsi ancora su questi temi e per migliorarci, laddove sarà necessario, ma oggi credo sia venuto il momento di dire, appunto, la parola definitiva su un provvedimento

dichiara improponibili per estraneità all’oggetto della discussione, ai sensi degli articoli 97 e 104 del Regolamento, gli ordini del giorno G8.100 e G39.101

Il vice ministro Oliviero, ambendo alla carica di Ministro, ovviamente si lancia in previsioni di modifiche normative.

Ma fate un decreto, lo prendete e diventa subito legge, punto. State rimpallando una cosa che qui dentro è stata inserita correttamente, è andata alla Camera, dove è stata tolta. Adesso l’emendamento viene trasformato in ordine del giorno e il vice Ministro si lancia dichiarando che sarà Ministro, vedendo come è stato gestito questo provvedimento, mi sa che si sta arrischiando la sua carriera politica in maniera eccessiva.

puntualizzare che questo emendamento è volto a inserire la clausola di invarianza degli oneri finanziari. Per l’ennesima volta chiediamo che si tenga conto del fatto che il comparto agricolo è sempre il solito bancomat utilizzato dal Governo. Dal comparto agricolo, infatti, vengono poi spostati dei fondi che potrebbero essere utilizzati per altre partite

in un momento di crisi, è opportuno evitare di penalizzare non solo il comparto, ma tutti i cittadini italiani. Quindi, chiediamo al Governo di rivedere una posizione diversa in confronto a quella avuta finora finora e di sopprimere l’ultimo periodo del comma 4, di sostituirlo con la clausola di invarianza finanziaria o, in mancanza, di prevedere

d’accordo con il Governo, è in ordine alle disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti. Che cosa significa?

avvenuti, le quali, per una ragione qualsiasi, rimangono giacenti presso le tesorerie provinciali dello Stato. Ho predisposto l’emendamento

di trasformarlo in un ordine del giorno, che potrebbe essere accolto nella misura in cui presentasse l’indicazione «a valutare la possibilità di» porre in essere da parte del Governo quanto

di queste indennità si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Scrivere, allora (come si fa nell’emendamento 9.1, sottoscritto anche dai colleghi Amidei e Scoma del Gruppo Forza Italia),

procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell’esistenza degli importi giacenti. Trascorsi centottanta giorni - quindi con un termine Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli.

a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare, il quale deve essere versato al CONOE, uno dei cosiddetti consorzi obbligatori. Il tema dei consorzi obbligatori è assolutamente delicato delicato e dovevamo affrontarlo al momento dell’approvazione del collegato ambientale. In quella sede, però, la valutazione del Parlamento fu di stralciare l’intera materia essendoci oggi assoluta consapevolezza che la questione dei consorzi è meritevole di un riordino complessivo. Tra l’altro, su questo argomento c’è una serie di pronunciamenti in sede europea

che,_ con l’ordine del giorno G10.100, sottoponiamo all’Aula la necessità di procedere a un riordino complessivo della disciplina dei consorzi

economico. Proprio per queste ragioni chiediamo un preciso intervento del Governo; anzi, auspico che risponda a questo mio intervento

proprio per alcune considerazioni che ha svolto precedentemente il collega Marinello. È giusto che in una fase iniziale dei prodotti cosiddetti secondari,

e assumono un loro valore intrinseco. Pertanto, far pagare ulteriormente un prodotto che non è più un rifiuto - come dicevo prima - ma ha un suo valore intrinseco, diventa contraddittorio. Per cui, questo è un provvedimento che dovrebbe avere una temporalità di uno o due anni e che poi dovrebbe essere superato da logiche di mercato. Per queste ragioni, abbiamo presentato emendamenti soppressivi in tal senso.

Non dimentichiamo che, proprio per il settore lattiero-caseario, stiamo lavorando per una forte aggregazione

Sottolineo che stiamo parlando di associazioni di categoria maggiormente rappresentative, non di aziende singole. Naturalmente, all’interno delle associazioni di categoria molte volte vi sono anche soggetti piccoli, che però si aggregano e che quindi, come tali, poi sono beneficiari. La nostra logica è aggregativa: non è volta a favorire i grandi, ma a spingere tutti i soggetti a trovare forme aggregative tali da poter poi essere rappresentativi e quindi anche affrontare le crisi di mercato come quella attuale.

Presidente, ritengo che l’articolo 15 sia il più importante di tutti quelli che abbiamo trattato fino ad adesso.

degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole premesso che il Governo necessita di dodici mesi dall’entrata in vigore di questo testo

un lavoro molto proficuo ed anche responsabile, conoscendo la delicatezza della materia che stiamo trattando.

Se me ne dà la possibilità, signor Presidente, vorrei leggere a chi è poco attento a questa materia, la lettera del secondo comma, che recita esattamente quanto segue: «revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

Mi sorge un dubbio, perché, esattamente sei mesi fa, è stato nominato il consiglio di amministrazione di ISMEA, che è uno degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e, guarda caso, dopo pochi mesi esce il consiglio di amministrazione ed entra trionfante un commissario, poi si nomina il commissario di AGEA e si fa fuori l’indomani mattina. Possiamo chiedervi quando finirete di fare queste manfrine? Gli enti vigilati rappresentano, in termini di spesa,

dei sacrifici dei nostri contribuenti, degli italiani.

vigenti richiamando articoli di legge, quindi in maniera particolarmente criptica, però, in realtà, essa è connessa ad un percorso molto lineare che è stato compiuto di accorpamento

favorevole

quanto era stato approvato dal Senato in prima lettura: si tratta di interventi che servono davvero all’agricoltura, come la modernizzazione della rete dei mercati all’ingrosso, lo sviluppo dei poli logistici per il potenziamento dell’intermodalità

articolo indicava una certa ambizione e la volontà di intervenire là dove si possono potenziare le possibilità delle aziende agricole italiane

Per questa pianificazione si autorizzano le organizzazioni dei produttori (OP), che si stanno consorziando in AOP, delineando quindi quel meccanismo di concentrazione che il Vice Ministro faceva presente poc’anzi,

la produzione di latte, in modo tale che questa possa gestirne al meglio la produzione e la commercializzazione, bensì si consente alle OP di accedere alla banca nazionale dell’anagrafe zootecnica

la trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento 22.1. Stiamo parlando di mense scolastiche. Comprendo le difficoltà che il Governo ha a far passare in sede europea

un ulteriore contributo, che rimetto al Governo, nella persona del vice ministro Olivero. Credo che, per raggiungere questi obiettivi, sui quali mi sembra ci sia ormai una sensibilità diffusa, e per eludere nella maniera più legale possibile le stringenti prescrizioni europee, si potrebbe adottare la formula delle sollecitazioni a favorire procedure di gara nelle quali l’elemento del chilometro zero e del biologico diventino requisito di premialità.

non solo a promuovere la nostra economia, ma anche un principio di salute alimentare condiviso ormai da tutto il mondo della scienza. Credo che, se noi provassimo a forzare la mano negli impianti di procedura di gara con questa indicazione, potremmo ottenere il rispetto delle norme europee, ma anche provare ad invertire una rotta.

Noi, però, in Commissione agricoltura stiamo già discutendo di un provvedimento organico e completo che affronta questi temi e, quindi, non è un tema rispetto al quale la Commissione sia distratta. Anzi, siamo a un punto molto avanzato. Sulla valutazione dell’accoglimento mi rimetto al Governo. L’intenzione e la valutazione complessivamente sono positive; tuttavia, ci dica il Governo se intende accogliere questa anticipazione.

abbiamo già messo alcuni tasselli nei provvedimenti di legge approvati recentemente. In particolare, segnalo, oltre alla buona scuola, nel quale si inseriva l’elemento per quanto riguarda le mense scolastiche,

compatibilmente con le normative europee. Accolgo l’osservazione del senatore Stefano, che è molto giusta, perché la compatibilità con le norme europee sta nell’inserire

Il tutto è quindi alquanto strano e, in alcuni casi, inquietante. Non si riesce a capire perché si debba mantenere una definizione che lascia pensare a ben altro rispetto a problemi di natura fiscale.

Presidente, quanto hanno appena detto il senatore Malan e precedentemente il senatore Ruvolo è degno di assoluta attenzione e considerazione. Vede, signor Presidente, qui ci troviamo di fronte a un paradosso. Il relatore, relatore, che ha facoltà di presentare emendamenti in qualsiasi momento dell’iter di esame di un provvedimento, si limita invece alla presentazione di un ordine del giorno;

questi dovrebbero essere considerati e diventare parte integrante del provvedimento normativo. Invece cosa accade? Accade che il Governo, per sua negligenza, ha lasciato macerare il provvedimento, non come il luppolo o l’orzo per la birra, ma per utilizzarlo per utilizzarlo poi come elemento di ricatto nei confronti del settore stesso. Adesso, arrivando al pettine il nodo, ci troviamo con ci troviamo con il settore che fa presente al Governo che ci sono delle incongruenze. Stiamo parlando della produzione della birra, dei microbirrifici, della grande distribuzione e degli annessi e connessi. E il Governo cosa fa? Non tiene conto di questi elementi. Il relatore si limita, con un ordine del giorno, a impegnare il Governo neanche in maniera definitiva, ma a “valutare l’opportunità di”, con la classica formula che assimila il voto che dopo faremo, purtroppo, a quello scritto sulla carta del burro (per non dire peggio). Se ci deve essere una presa di coscienza, questa deve essere seria. Quindi si sopprima l’articolo oppure il Governo dia la sua disponibilità all’approvazione degli emendamenti successivi, che tengono conto dei rilievi fatti dal settore stesso e da chi produce,

Stia attento ovviamente il Vice Ministro a non prendersi troppe responsabilità nel dare un parere magari favorevole agli emendamenti, perché la sua carriera politica ne sarebbe messa a rischio.

Ciononostante, credo sia opportuno accogliere gli ordini del giorno in questa direzione, essendo materia che per la prima volta viene affrontata e rispetto alla quale è necessario procedere anche il Governo dovrà monitorare nei prossimi mesi quali sono le risultanze della norma introdotta ed, eventualmente, apporre correttivi o elementi migliorativi nel testo per gli anni a venire. È un settore, come è stato rimarcato nel dibattito generale da diversi

per noi oggi, anche rispettosi del lavoro svolto dai colleghi della Camera dei deputati, è quella di accogliere questo testo, però, naturalmente, come Governo, di monitorarne l’efficacia al fine di poterne eventualmente andarla a migliorare

precluderebbe di aprire gli habitat naturali alla fauna selvatica locale. Si tratta di un ordine del giorno e di un impegno sul quale tutte le organizzazioni del settore hanno espresso

Esprimo parere contrario sull’emendamento 39.1. Per quanto riguarda l’ordine del giorno G39.100, il parere è favorevole, anche se il Governo aveva chiesto una piccola riformulazione, che prego

rimetto al Governo. al proponente, senatore Stefano, è di espungere, nell’impegno al Governo, l’inciso «quali la trota fario e la trota iridea».

da parte delle Camere, è opportuno che siano i soggetti preposti di natura tecnica a valutare quale siano le specie che creano pregiudizio agli habitat naturali

dalla Camera, introduce indubbiamente un disallineamento della norma sul tema degli sfalci e delle potature tra la direttiva n. 98 del 2008 sui rifiuti e il decreto legislativo n. 152 del 2006, che comunque continua a classificare questa tipologia di rifiuti come rifiuti urbani. Stiamo parlando di un milione e mezzo di tonnellate di sfalci e potature che vengono attualmente differenziate, avviate agli impianti di compostaggio e, attraverso un processo di trattamento biologico, in un percorso di recupero di materia; si tratta di un processo che comunque ne garantisce la fase di igienizzazione, l’abbattimento dei patogeni e ovviamente la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria.

essere veramente preso in seria considerazione quanto io e il senatore Piccoli facciamo presente. È assurdo pensare che un prodotto nel caso di specie un sottoprodotto - non possa essere considerato tale nel momento in cui il trattamento meccanico avvenga sul posto di produzione.

e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di circoscrivere la portata normativa dell’articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali.

Pertanto gli agricoltori (oggi parliamo di agricoltori, ma per la verità non solo di loro, perché questi materiali possono derivare anche da attività non propriamente agricole)

di difficoltà che attraversa il settore, per la concorrenza internazionale, per le mille ragioni di cui sappiamo, per le modifiche nella politica agricola comunitaria e così via.

perché non si estenda tale buon senso al materiale trattato meccanicamente sul posto di produzione, cioè in un modo anche virtuoso. Francamente è difficile per noi che abbiamo una certa abitudine alle procedure legislative, figuriamoci per l’agricoltore e per l’operatore che si trovano a fare un lavoro assai più pratico di quello che ci troviamo a fare noi. Possibile che non si possano si possano mantenere queste caratteristiche con questo trattamento e con queste previsioni legislative anche nel caso di prodotti che vengono trattati meccanicamente sul posto di produzione? Francamente è difficile capirlo. Anche l’emendamento 41.2 meritava una sua attenzione. Anziché circoscrivere in modo eccessivo e, francamente, poco comprensibile l’appli

materiale proveniente da lavori agricoli e forestali. Quando si dice che si vogliono semplificare le leggi, bisogna pensarci tutti i giorni; non bisogna aspettare che arrivi la legge di semplificazione, che di solito è di complicazione.

spianare la strada a coloro che vogliono lavorare nel nostro Paese, specialmente in un settore difficile come l’agricoltura. Non dovrebbe creare ostacoli artificiali e cambiare le norme a ogni giro di calendario. Ecco perché chiederei a tutti il voto favorevole e, più in generale, un atteggiamento di maggiore lungimiranza nel fare le leggi. Non dobbiamo fare le leggi perché abbiamo una scadenza o dobbiamo andare a pranzo. Le leggi devono essere a favore dei settori di cui ci occupiamo.

il Governoa monitorare e valutare gli effetti applicativi dell’articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di circoscrivere la portata normativa dell’articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali.

ai servizi sociali e poi alle cure di una famiglia. Nel frattempo, nei confronti dei suoi genitori naturali, a ragione della loro età anagrafica - un’età effettivamente avanzata in maniera inconsueta rispetto a quella in cui normalmente si concepiscono i figli e a causa della quale, nel 2010, quando la bimba nacque, si scatenò anche una particolare attenzione mediatica

Ciò che colpisce è che, alla base di queste sentenze c’era la presunzione di un atto di abbandono da parte dei genitori stessi nei confronti della bimba.

Attraverso un’istanza di revoca, la settimana scorsa la stessa Corte di cassazione ha determinato invece che l’adottabilità non può essere sentenziata e che quella bambina, anche alla luce delle verifiche ulteriormente fatte sulle caratteristiche sociali, culturali, morali dei genitori, può essere riaffidata alle cure della famiglia stessa, rimandando la sentenza adottata dalla stessa Corte di cassazione all’esame della Corte d’appello di Torino. Naturalmente io non ho né gli strumenti giuridici né quelli di formazione psicologica o sociologica per esprimere una valutazione compiuta nel merito. Certamente, in questa vicenda lasciano sconcertati ed esterrefatti

Queste distonie della giurisprudenza producono un danno, prima di tutto nei confronti di un minore, che comunque oggi ha sei anni e per sei anni non ha potuto avere una famiglia. Quindi, mi auguro che questo ci possa fare da lezione. (Misto-Idv). Gentili colleghi, tutti noi conosciamo il significato della parola «dono»: è ciò che si dà o si riceve senza niente in cambio. Proprio in questa legislatura abbiamo dedicato una giornata, il 4 ottobre, al dono per offrire a tutti noi cittadini l’opportunità di riflettere sul contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nelle quali i valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano un’espressione degna di essere riconosciuta e promossa. Per questo trovo necessario porre l’accento su una vicenda che poco ha da condividere con questa alta definizione di dono. È la vicenda dei defibrillatori “donati” dai consiglieri regionali toscani del Movimento 5 Stelle ad alcune istituzioni scolastiche, Comuni e associazioni del territorio, acquistati devolvendo gettoni di presenza. Si tratta di un’iniziativa ammirevole e rispettabilissima, se non fosse che i consiglieri pentastellati hanno preteso che insieme al defibrillatore fosse accettato dai destinatari del dono anche un cartello di spiegazioni con il logo del partito in bella evidenza. Senza il cartello e il logo, niente dono. Si capisce che molte scuole, che avrebbero volentieri accettato un oggetto così utile, sono state costrette a declinare l’offerta perché in un luogo pubblico, specialmente in una scuola, è del tutto inappropriato esporre simboli di partito. Anzi, tenuto conto della normativa sulla propaganda elettorale, i dirigenti scolastici sarebbero potuti incorrere in sanzioni. Sarebbe bene, quindi, che i parlamentari del Movimento 5 Stelle spiegassero ai loro colleghi a livello regionale la differenza tra dono e ricatto ed evitassero di fare della solidarietà una bieca propaganda politica al limite della compravendita dei voti.

Signor Presidente, la Sicilia versa in emergenza rifiuti da mesi, anzi anni, a causa dell’assoluto pressappochismo del governo Crocetta, che si è mostrato incapace di affrontare con una seria progettualità la questione rifiuti. La situazione è precipitata da fine maggio, quando il Governo regionale ha esaurito le deroghe a disposizione per affrontare l’ennesima emergenza annunciata, tra l’altro in una Regione con il più basso tasso di raccolta differenziata e un sistema di discariche praticamente al collasso, molte delle quali private. Succede così che lo scorso 7 giugno la Giunta Crocetta, di concerto con il Governo Renzi, trova l’ennesima soluzione tampone. La soluzione di Crocetta e del suo assessore al ramo, Vania Contrafatto, è quella di far conferire i Comuni di mezza Sicilia nella discarica di Lentini, in Provincia di Siracusa, costringendo gli amministratori locali a fare i conti con viaggi in alcuni casi anche di 500 chilometri (come nel caso di Marsala: oltre 250 chilometri per l’andata e altrettanti per il ritorno degli autocompattatori) per conferire i rifiuti in discarica. Come se tutto ciò non bastasse, da alcuni giorni è avvenuto l’impensabile: i Comuni hanno fatto partire i compattatori carichi di rifiuti che, dopo aver attraversato l’sola, hanno trovato i cancelli della discarica chiusi chiusi e sono dovuti tornare indietro. La discarica di Lentini, intanto, a meno di un mese dall’ordinanza del presidente Crocetta, non ha più dove mettere i rifiuti e li sta mandando in Bulgaria, a costi enormi per la collettività. Tutto questo sta avvenendo in mezza Sicilia: da Carini a Marsala, da Porto Empedocle a Mazara del Vallo. A Carini, ad esempio, il sindaco si ritrova a combattere contemporaneamente su due fronti: da una parte quello del personale ATO insoddisfatto e frustrato, dall’altra quello delle discariche costosissime e che si chiudono a intermittenza. In Provincia di Trapani, i Comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano hanno depositato un esposto al procuratore di Marsala, perché in questo caos si rischia chiaramente l’emergenza igienico-sanitaria. Sapete come si è difeso il Governatore siciliano? Ha detto che «c’è una parte dell’assessorato rifiuti, non certo l’assessore, che lavora contro il mio Governo per non risolvere l’emergenza», come se a guidare l’amministrazione regionale non fosse il presidente Crocetta e quella «parte dell’assessorato» che rema contro non fosse sotto la sua diretta responsabilità. In una Regione amministrata da nessuno, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e su questo il Partito Democratico dovrebbe fare una serissima riflessione.